grazie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

di questo disegno di legge, della cosiddetta autonomia. Si tratta, infatti, di un disegno di legge che viola il diritto di uguaglianza e il principio di solidarietà che sono alla base della nostra Costituzione e della nostra democrazia. un disegno di legge che incide sui diritti fondamentali e li rende diseguali. Voi - Presidente, mi rivolgo per suo tramite ai parlamentari della destra - scardinate quello che di più importante abbiamo, per cui tutti, ovunque risiedano, abbiano la stessa parità di accesso ai beni comuni essenziali, come la sanità e la scuola. Già oggi ci sono diseguaglianze e divari insostenibili, ma voi adesso li allargate, li certificate per legge e li rendete definitivi e irrecuperabili, con conseguenze che saranno drammatiche sulle vite dei cittadini e che condanneranno interi territori alla marginalità e allo spopolamento. L'istruzione è quella che permette a ogni bambino di emanciparsi e crescere libero. Per questo è così importante il carattere universale e nazionale dell'istruzione, che è una delle conquiste fondamentali della nostra Costituzione (mi riferisco agli articoli 33 e 34). Voi, invece, in aperto contrasto con la Costituzione, come ribadito da numerose sentenze della Consulta, volete permettere di attribuire ad una Regione la competenza esclusiva sull'istruzione. E questo è gravissimo, perché mette a rischio - un rischio mortale - le basi del diritto allo studio, ciò che, tra mille difficoltà, la nostra Costituzione vuole che sia la scuola, cioè scuola inclusiva, aperta a tutti, garante dei diritti di tutti, obbligatoria e gratuita, dove c'è uguale trattamento degli alunni, dove la selezione e l'assunzione dei docenti sono uguali in tutto il Paese dove i capaci e i meritevoli, anche se privi di mezzi economici, hanno il diritto di andare avanti sostenuti dallo Stato. *(Applausi)*. che include chi è più debole, che non lascia indietro nessuno, che contrasta l'abbandono e l'insuccesso scolastico, che contrasta la povertà educativa, che spesso è tutt'uno con la povertà sociale. Voi colpite tutto questo, perché scardinate il principio costituzionale della competenza esclusiva dello Stato, che è alla base di un sistema di istruzione universale ed unitario. E sapete chi ne farà le spese? Voi la risposta la conoscete perfettamente. A farne le spese saranno le fasce sociali più deboli, i territori più deboli, le aree interne, perché l'istruzione è decisiva per lo sviluppo dei sistemi locali. A farne le spese saranno le ragazze e i ragazzi delle famiglie in difficoltà, i figli dei lavoratori poveri. Impedirete loro di avere opportunità al pari degli altri, quelle che la Costituzione assegna a tutti. Noi diciamo "no" a questo scempio, a questo tradimento, che voi fate, della Costituzione e dell'identità culturale del Paese. Volete ridurre l'Italia a tante piccole patrie senza destino. Invece, abbiamo bisogno di un'Italia più unita e più coesa. Questo è il significato dei nostri emendamenti e per tutto questo continueremo a dare battaglia.

Porto l'enfasi sul trasferimento delle funzioni, in particolare in tema di tutela ambientale, di cui agli articoli 9 e 41 della Costituzione. Appare veramente pericoloso, infatti, delegare funzioni in questa materia, perché la gestione statale la risorsa ambientale non può essere ristretta nell'ambito dei confini amministrativi di una Regione. Quando si parla di allocazione di risorse, bisogna pensare anche all'utilizzo delle risorse presenti, quindi allo sfruttamento dell'ecosistema e del capitale naturale, che è patrimonio comune, quindi italiano e non meramente regionale. E le ricadute dei danni all'ambiente pesano su tutti.

perché fa emergere un nodo importante e cioè quello delle cosiddette competenze concorrenti, sulle quali i proponenti - chiederei al collega

la suddivisione delle competenze concorrenti fra Stato e Regioni oggi rischia di aumentare il quadro della confusione, della burocrazia, della ridondanza e della inefficacia.

Tutto questo problema, però, sarebbe stato risolto se la famosa riforma Renzi-Boschi fosse stata resa operativa, perché questo tema era stato affrontato e risolto con la riforma approvata due legislature approvata due legislature fa e che anche alcuni dei proponenti di questo emendamento avevano fortemente contrastato. rivolgo ai colleghi del Partito Democratico e ai colleghi del MoVimento 5 Stelle che voteranno questo emendamento e anche ai colleghi della destra che condividono questa posizione ma non lo possono dire: se quella normativa fosse stata approvata, ci saremmo risparmiati tutto questo e sicuramente ci saremmo risparmiati questa legge Calderoli. Magari vi servirà a futura memoria.

non difendevano le scelte di procedura e le priorità di questo disegno di legge, ma facevano una sorta di ricostruzione, naturalmente parziale e propagandistica, sul concetto di autonomia differenziata, su chi la voleva e chi non la voleva. Io ieri mi sono chiesto per quale ragione ragione nessuno di coloro che è intervenuto ha difeso le procedure presenti nel provvedimento. Il disegno di legge non è stato difeso neanche dal Ministro. Allora per quale motivo si sceglie prima di fare le intese e poi di definire i LEP? Per quale motivo si sceglie di fare prima le intese e non di trovare le risorse per i LEP e poi di attuare i livelli essenziali delle prestazioni? Perché non si decide prima di ridurre le diseguaglianze e i divari territoriali e poi di attivare le intese? Sono due modalità diverse di attuazione dell'autonomia differenziata, ma che fanno grande differenza non solo sul lato dell'uguaglianza, ma anche sul lato dell'incentivo

vengono posposte perché tutta questa impostazione nasce dall'idea che se mai si dovessero avviare compensazioni nei confronti dei *loser*, dei perdenti dell'autonomia, questo sarà fatto dopo. che effettivamente crea disuguaglianza, divari e spacca il Paese. Se così non fosse dovremmo votare positivamente su questi emendamenti. Che problema c'è? Se è indifferente fare prima i LEP e dopo le

dell'autonomia differenziata di anni passati, peraltro con diverse mistificazioni? Cos'è che nascondete? Cos'è che non potete dire? Il voto su questi emendamenti può rivelare una forma di verità.

Signor Presidente, nel testo che ci è stato distribuito immagino vi sia un refuso - lo dico agli Uffici, visto che siamo in sede legiferante - perché

però lo vorrei chiedere per precisione, perché diversamente rischiamo un problema in sede di approvazione.

Presidente, questi emendamenti in realtà chiedono tutti una cosa, cioè che prima di chiedere l'autonomia su più materie sia richiesta una qualche motivazione. Questo noi l'abbiamo detto anche negli interventi che abbiamo fatto in Aula. Chiediamo come si pensi con questo provvedimento di attribuire alle Regioni che ne fanno richiesta 23 materie, da cui derivano 500 funzioni, dove c'è praticamente di tutto, dall'energia alla ricerca, dai contratti dei medici ai contratti degli insegnanti, non tenendo conto del fatto che c'è stata anche una commissione, istituita al Ministero degli affari regionali negli anni scorsi, che di fatto ha dimostrato che dall'attribuzione di più autonomia su alcune materie non deriva né un vantaggio chiaro dal punto di vista economico, né un vantaggio dal punto di vista burocratico. burocratico. Quindi, chiediamo ancora una volta alla maggioranza di riflettere e valutare l'opportunità di votare favorevolmente questi emendamenti.

è diretto a escludere dal possibile riconoscimento di ulteriori e particolari forme di autonomia alle Regioni le materie di legislazione esclusiva statale, come le norme generali dell'istruzione, e alcune delle materie di legislazione concorrente, per le quali una ulteriore devoluzione comporterebbe - a nostro avviso - una totale disarticolazione dei diritti fondamentali delle persone e finanche lo sviluppo economico unitario del Paese. Questa proposta in particolare nasce anche sulla base di una mobilitazione che c'è stata nel corso degli ultimi mesi nel nostro Paese. Noi facciamo nostro, come Alleanza Verdi e Sinistra, ma immagino assieme alle altre opposizioni, l'appello delle principali organizzazioni sindacali italiane (ad esempio, la CGIL del comparto istruzione e ricerca), e con esse anche di tutte le reti studentesche e le reti degli insegnanti, chiedono la salvaguardia del carattere unitario e nazionale del nostro sistema pubblico di istruzione. Secondo noi, è chiarissimo che, se

fondamenti intangibili - secondo noi - su cui si costituiscono la cittadinanza, la libertà, l'unità del nostro Paese e della nostra comunità. È evidente che siamo molto preoccupati dal fatto che eventuali leggi regionali potrebbero disciplinare l'istituzione di ruoli del personale della scuola, addirittura la stipulazione di contratti collettivi regionali e gabbie salariali (con devastanti conseguenze sulla tenuta delle finalità nazionali dell'ordinamento scolastico), il trattamento economico dei docenti, degli ATA e del personale, la mobilità territoriale, la valenza dei concorsi. Insomma, il rischio reale è di sbaragliare il sistema di istruzione così come l'abbiamo conosciuto e anche di mettere profondamente a rischio l'autonomia scolastica così come l'abbiamo conosciuta. Pensiamo che su questo punto si giochi davvero un pezzo rilevantissimo del futuro di questo Paese. Siccome pensiamo che la scuola sia la principale missione alla quale tutti noi dovremmo guardare come fondamento della Repubblica, riteniamo che l'approvazione di questo emendamento ci farebbe evitare un tale rischio. Lo dico al ministro Calderoli: ieri l'ho ascoltata, ha detto delle cose su questo mi dispiace, signor Ministro, perché quelle sue parole non possono rassicurarmi. Credo che il sistema istruzione nazionale sia profondamente a rischio se va avanti il progetto dell'autonomia differenziata e, almeno su questo punto, quello della tenuta della scuola pubblica di questo Paese, davvero vi chiedo di fermarvi.

da parte di una Regione, della stretta di un'intesa su determinate competenze sia motivata e vi sia la dimostrazione che, affidando quelle competenze a quella determinata Regione, i servizi e la qualità della vita dei cittadini ne troveranno un miglioramento. Questa è soltanto una richiesta di ragionevolezza che voi continuate a bocciare e che in questo testo non è contenuta. Ma lo spregio delle regole, Presidente, è diventato ormai il *modus operandi* di questa maggioranza e di questo Governo. A me non basta che si sia rinviato il voto definitivo su questo testo al prossimo martedì. Quello che è andato in scena in quest'Aula, purtroppo, è il completo spregio delle regole. Questo fascicolo sarebbe stato molto più nutrito di emendamenti, Presidente, come lei ben sa, se in Commissione bilancio non fosse stato utilizzato in maniera indiscriminata l'articolo 81, salvo poi rifilare un emendamento molto simile a quelli che sono stati respinti in Commissione da parte della maggioranza. Mi si dice che far rivivere quegli emendamenti sarebbe stato troppo complicato per via del Regolamento. Eppure, il Regolamento non conta niente per questa maggioranza, quando ieri, nella Commissione della Camera, dopo un voto fatto, poiché non era stato raggiunto il risultato da voi auspicato, si è ripetuto il voto. *(Applausi)*. Il Regolamento non conta niente, quando volete; lo invocate soltanto a convenienza.

che vede il parere favorevole del Governo e verrà quindi approvato, toglie dall'elenco delle materie che possono essere oggetto di devoluzione a una o più Regioni la lettera *a)*, e in particolare l'organizzazione della giustizia di pace. Approvando questo emendamento, emendamento, il disegno di legge Calderoli non ripeterà più in maniera pedissequa l'elenco delle materie di cui all'articolo 116, ma escluderà l'organizzazione della giustizia di pace. Ora io vorrei che il Ministro o i relatori spiegassero all'Assemblea per quale motivo escludono l'organizzazione della giustizia di pace e non invece

di trasporto, porti e quant'altro. Onorevoli colleghi, ci avete detto in Commissione che non era possibile

in Aula voi stessi escludete una materia. Noi non voteremo contro questa esclusione, ma vi chiediamo di spiegare per quale motivo

avessero la competenza esclusiva a disciplinare la produzione e la distribuzione nazionale dell'energia? Ma vi sembra una cosa possibile? Vi sembra una cosa seria? Bene, voi questa norma la conservate. Lo stesso vale - lo ripeto - per istruzione, sanità e trasporti. Mi fermo qui e spero che ci sia una risposta.

Annullo la votazione. Presidente, vorrei intervenire su questo emendamento col quale noi semplicemente chiediamo che, nella determinazione dei costi e dei fabbisogni *standard*, si tenga conto delle specificità territoriali e degli svantaggi derivanti dell'insularità. Esiste da poco, da meno di due anni, una norma costituzionale, l'articolo 119, comma 6, che riconosce le peculiarità delle isole e promuove le misure necessarie per rimuovere gli svantaggi derivanti dell'insularità. Finora, in questo provvedimento non avete voluto riconoscere che la determinazione dei LEP tenesse conto di questi svantaggi e non avete accettato che la Commissione parlamentare per il istituita da questo Parlamento, esprimesse pareri nelle procedure per l'adozione delle intese, né nell'aggiornamento dei LEP (è un emendamento appena bocciato). Il Governo non ha finanziato il Fondo per la rimozione degli svantaggi derivanti dall'insularità, istituito con la scorsa legge di bilancio su proposta del Partito Democratico. Insomma, non si tiene conto dell'insularità, se non con qualche parola inserita in questo provvedimento, ma questa mattina il ministro Calderoli è venuto in audizione presso la Commissione parlamentare

perché non approvare questa misura? Perché non approvare questo emendamento? *(Applausi)*. Perché non scriverlo chiaramente in maniera vincolante nella legge? Altrimenti, l'insularità è una parola che usate, perché voi - come noi - avete le elezioni in Sardegna, perché la Sicilia ugualmente ha lo stesso problema, ma sarà una parola vuota. Chiedo pertanto di cambiare questo parere, di tener conto di questo principio e di ancorarlo a una norma legislativa che abbia una qualche certezza.

che sostanzialmente ricorda l'esistenza di un articolo della Costituzione, cioè il 119: se questo però è necessario, penso che debba essere fatto allora per tutti gli articoli, ai sensi di un corrispondente articolo della Costituzione. Mi meraviglierebbe

Si è anche cercato di incolpare in qualche modo il MoVimento 5 Stelle, che allora non era neanche nella mente degli dei. Tutti qui, a chiacchiere, siamo d'accordo che quella modifica del Titolo V del 2001 sia stata un errore: è stata scritta male e sarebbe da modificare. Vi è stata servita sul piatto d'argento la possibilità di modificarla, magari davvero tutti insieme: insieme: c'è stata una legge di iniziativa popolare che è sbarcata in quest'Aula, ma voi avete umiliato la volontà popolare, mettendola all'ordine del giorno dopo la legge ordinaria. Allora, ameno un pezzetto insieme lo vogliamo fare? Questo ordine del giorno chiede un impegno ad

vogliano venti sistemi educativi e formativi diversi nella nostra Nazione, con il rischio di creare venti culture diverse e contrapposte all'interno del nostro Paese. Ripensateci e almeno prendete l'impegno a estrapolare la cultura e l'istruzione

*Al comma 1, in fine, sostituire le parole da:* «coerenti con gli obiettivi programmati» *fino alla fine del comma con le seguenti:* «volte ad assicurare i medesimi livelli essenziali delle prestazioni sull'intero territorio nazionale, ivi comprese le regioni che non hanno sottoscritto le intese, al fine di scongiurare disparità di trattamento tra regioni, coerentemente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica e con gli equilibri di bilancio, nel rispetto dell'articolo 9 della presente legge e della lettera *d)* del comma 793 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022,

L'emendamento 4.203, depositato per l'Assemblea l'11 gennaio, alla scadenza della presentazione degli emendamenti, ha avuto una riformulazione questa mattina da parte del Governo, dopo una settimana, e non ci sono stati consentiti neanche dieci minuti per poter valutare quella riformulazione. Per tale ragione abbiamo chiesto una riunione della Conferenza dei Capigruppo informale per gestire i passaggi successivi. La cosa più grave è che non troverete in questo fascicolo emendativo

irrispettosa non delle prerogative della maggioranza e dell'opposizione, ma dei singoli parlamentari, che sono prerogative che tutti noi assieme dovremmo cercare di tutelare il più possibile. Oggi infatti non troviamo testi

Il combinato disposto di questa previsione e dal fatto che discutiamo un disegno di legge che in modo, a nostro avviso, surrettizio, è collegato alla legge di bilancio, preclude la possibilità preclude la possibilità emendativa. Ritengo che su tale questione dovremmo impegnarci tutti per fare chiarezza una volta per tutte. Le regole del gioco devono essere identiche per tutti.

un piccolo rimedio, un pannicello caldo di fronte al vero problema di come questo disegno di legge vuole normale l'attuazione dell'autonomia differenziata. Il vero problema è che vuole farlo a saldi invariati e questo è assolutamente impensabile, se non si vuole distruggere completamente la coesione del Paese. *(Applausi)*. Pensare di attuare l'autonomia senza risorse è una presa in giro per gli elettori delle elezioni europee, ma non può passare in quest'Aula, perché abbiamo sufficiente esperienza per capire che l'obiettivo è soltanto quello, poter sventolare l'approvazione dell'autonomia differenziata prima delle elezioni europee,

stiamo parlando di una straordinaria operazione di mistificazione comunicativa, perché, nella suddivisione delle parti in commedia che la maggioranza si è data, la Lega si

non preoccupatevi, perché le cose che daremo al Nord le garantiremo anche a tutto il Paese. Tutto ciò nel silenzio di Forza Italia, che evidentemente assiste senza poter più dire nulla. In questo scenario, l'emendamento 4.203 afferma un elemento paradossale, signor Presidente, garantiamo tutto a tutti e diamo più soldi ad invarianza di spesa. Se non è una presa in giro questa, non so che cosa lo sia. *(Applausi)*. Garantiamo tutto a tutti e diamo soldi a tutti ad invarianza di spesa. Capisco che, nella comunicazione sincopata in cui la politica oggi vive, tutto quello che diciamo alle ore 11 del mattino venga bruciato alle ore 18 della sera e ciascuno debba raccontare la propria parte in commedia. però, stiamo approvando una legge e, proprio perché crediamo ancora nel valore della legge e nel valore della politica, non possiamo votare questa presa in giro. Presidente, con la riformulazione presentata dal relatore e accolta del Governo si introduce un pericoloso precedente,

ha creato una disparità di trattamento tra gli emendamenti presentati dalle opposizioni e quelli che oggi servono in quest'Aula per mascherare le divisioni della maggioranza e fare in modo che questo manifesto arrivi a compimento. una violazione delle prerogative non tanto di questo Parlamento, ma anche del lavoro della Commissione bilancio, perché è stato utilizzato quanto disposto dall'articolo 81 della Costituzione, non consentendo ai singoli parlamentari di venire a presentare in Aula emendamenti e discutere anche con la maggioranza delle regole fondamentali dentro le quali la cornice dei LEP avrebbe dovuto muoversi. Questo dibattito è durato tre mesi e fin qui ci è stato detto che dei LED se ne sarebbe occupata la Commissione e che tutto doveva avvenire a invarianza di spesa, che questo ha pregiudicato il lavoro del Parlamento e dell'intera maggioranza. Gli emendamenti hanno pari dignità, signor Presidente; non si possono stabilire quali tra quelli della maggioranza abbiano bisogno di una relazione tecnica per risolvere i problemi della maggioranza Gli emendamenti dovrebbero servire per migliorare un testo e garantire al Paese iniziative legislative corrette e appropriate. Questa operazione, signor Presidente, ovviamente non cambia nulla, perché la riformulazione di fatto sterilizza possibili effetti finanziari. Continuate cioè a vendere al Paese un manifesto che risulterà inattuabile e servirà a voi per portare a casa la presunta coesione di questa maggioranza, ma purtroppo sarà un prezzo caro che pagherà il Paese, perché mettete questo manifesto in contrapposizione con l'interesse nazionale. Se si vogliono ridurre i divari territoriali, si deve operare dentro un federalismo cooperativo, che metta al centro l'interesse nazionale e non gli egoismi particolari dei singoli territori. Giocate col fuoco, ampliando le disuguaglianze e creando un percorso inattuabile e pericoloso per aumentare i divari e non favorire nuovo sviluppo economico.

che bisogna tener conto non solo di quelli che faranno l'accordo, cioè delle Regioni che utilizzeranno l'autonomia differenziata, ma anche delle altre; dev'essere sostanzialmente alla pari, a costi invariati. Ma a chi volete darla a bere? Ieri sono intervenuto in discussione generale, dimostrando quanto grandi siano le disuguaglianze in questo Paese. Per ridurre le disuguaglianze bisogna spendere i quattrini. E allora smettete di fare la propaganda che avete già annunciato oggi sui giornali! Questo è il dato vero: avete voluto dare dare un dito negli occhi all'opposizione e a noi. Avete sbagliato e vi abbiamo chiesto di fermarvi. Ovviamente noi non ci fermeremo e andremo avanti, utilizzando tutti gli strumenti,

intervengo in dissenso dal mio Gruppo, ma con il consenso del mio Capogruppo, naturalmente perché la questione tecnica inerente a questo emendamento è stata spiegata, ossia l'abuso fatto in Commissione bilancio

...che state realizzando il sogno proibito della Lega Nord, ossia la secessione e il federalismo di fatto. E metterci una pezza come questa foglia di fico non servirà a poter guardare in faccia i vostri elettori del Meridione, al termine di questa giornata.

sinceramente rammaricato del fatto che, durante i nostri lavori in 1a Commissione, non abbiamo potuto esaminare e votare alcuni emendamenti, non soltanto dell'opposizione, ma anche della maggioranza,

su questa cosa vada avviata una riflessione, perché non si può privare il Parlamento della possibilità di esaminare provvedimenti che vanno nell'interesse generale, per motivi che molto spesso io personalmente, insieme a molti colleghi, ho dovuto constatare che apparissero contraddittori e a volte addirittura inspiegabili, se non del tutto infondati.

Credo di essere stato chiaro su questo punto, perché è davvero mortificante per tutto il Parlamento, ma in particolare per la 1a Commissione, dover soggiacere a questi *diktat*. Non si può andare avanti così. La prego di rappresentare questo mio punto di vista, che credo corrisponda a quello della grande maggioranza di quest'Assemblea. È ancora più mortificante per me, ma credo per tutta la maggioranza in quest'Aula,

È mortificante per la maggioranza - immagino anche per il senatore De Priamo e per la mia forza politica, che si è battuta moltissimo, come tutti sanno, affinché questo emendamento entrasse nel testo della legge - non poter realizzare oggi una convergenza unanime o quasi su questo tema. Infatti, se la logica non mi fa difetto, nel momento in cui forze politiche di opposizione affermano qui solennemente di aver presentato emendamenti uguali a questo, ciò significa che, se avessimo avuto la possibilità di confrontarci nel merito già in Commissione, probabilmente saremmo arrivati con questa

loro. Posso soltanto esprimere il mio rammarico e il mio dispiacere, perché questa è una legge che dev'essere scritta nel modo migliore possibile. Noi ci siamo adoperati in tale direzione. Se me lo consente, signor Presidente, concludo

ivi comprese le Regioni che non hanno sottoscritto le intese (e questo era un punto pregiudiziale per Fratelli d'Italia) «al fine di scongiurare disparità di trattamento tra Regioni», ma, fate bene attenzione, coerentemente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica e con gli equilibri di bilancio; non c'è scritto a invarianza di bilancio.

Credo sia l'unico intervento che farà il mio Gruppo, quindi la prego di essere generoso anche con noi, Non ci siamo mai stancati di spiegare che questo disegno di legge prevede l'invarianza finanziaria, perché è una norma procedimentale. Sarà in sede di intese che verranno trovate e stabilite le risorse e sarà questo Parlamento a votare la legge con la quale si finanzierà la devoluzione di determinate materie. Noi oggi stiamo stabilendo i criteri con cui questo dovrà avvenire. Non stiamo stabilendo come finanziare quell'ulteriore processo che oggi stiamo avviando.

non cerchiamo di mettere i carri davanti ai buoi e di confondere la questione. Per queste ragioni, voteremo a favore dell'emendamento

Poteva essere riformulato. La prossima volta - glielo dico, signor Ministro - attuerò un diverso atteggiamento: in Commissione non consentirò più di fare riformulazioni, perché,

Presidente, intervengo sull'ordine dei lavori - lo dico anche ai fini del computo del tempo - per porre una domanda alla Presidenza, nell'ambito dei cinque minuti che ho a disposizione ai sensi del Regolamento. Noi abbiamo ascoltato con grande attenzione l'intervento del presidente Balboni e ci sono due aspetti che questo intervento in Aula porta con sé. Un primo aspetto è sicuramente di natura politica. Non mi soffermo più di tanto, ma non sfugge a nessuno che un autorevole, oltre che stimato (almeno da chi le parla), ha chiaramente posto una censura politica nei confronti del Governo. Lo abbiamo sentito tutti: ha posto una questione di estrema rilevanza politica. Lo registriamo e non può, almeno dal nostro punto di vista, passare sotto silenzio. La seconda questione non è una questione banale. Il Presidente della 1a Commissione del Senato ha fatto rilevare che l'intervento odierno del Governo

Io potrei entrare anche nel merito e vorrei farlo per piccolo inciso, soltanto per spiegare perché noi non possiamo, anche se avremmo voluto farlo, sottoscrivere questo emendamento. L'emendamento originario diceva che originario diceva che «sono contestualmente incrementate le risorse volte ad assicurare i medesimi livelli essenziali delle prestazioni»: che sono contestualmente incrementate. L'intervento del Governo di oggi ha cambiato, come ho cercato di descrivere, le carte in tavola. Ora, però, si pone un problema anche procedurale, nel senso che la Commissione di merito, la 1a Commissione, ha licenziato il testo partendo dal presupposto che ci sarebbe stato un impianto di un certo tipo. Ora il Governo, con un *blitz* che è stato descritto anche dai colleghi in precedenza, modifica le carte in tavola. Il Presidente della 1a Commissione viene qui e ci dice

dal suo collega del MEF), che questa è la prima e l'ultima volta che succede una cosa di questo genere, perché non si possono né cambiare le carte in tavola né modificare le prerogative proprie degli organi interni al Senato. La Presidenza non può non porsi questo interrogativo, perché noi stiamo licenziando un testo su cui il Presidente della 1a Commissione ci dice che c'è stato un *vulnus* a danno della Commissione di merito, che è la Commissione che obbligatoriamente deve rendere un parere a tutti i provvedimenti di questa Camera. Se questo non è un elemento da sottolineare, io mi chiedo che cosa lo sia. In conclusione, se intendete procedere ulteriormente, anche rispetto a questa tematica, se la Presidenza non riterrà di svolgere un approfondimento di carattere procedurale, alla luce dei rilievi fatti dal presidente Balboni in questa sede, è di tutta evidenza che si è aperto un problema politico,

questo dibattito interrotto da due Presidenti di Commissione, il presidente Balboni prima e il presidente Calandrini poi, ci impone una riflessione seria che, per quanto riguarda il Gruppo Partito Democratico, dovrà essere portata nella prossima Conferenza dei Capigruppo, perché questo dibattito non può finire così.

Se apprezziamo l'onestà intellettuale che in quest'Aula deve essere sempre anteposta ad ogni intervento, presidente Balboni, senza un atto conseguente il suo sforzo intellettuale rischia di essere un vano tentativo di salvare la coscienza

dalla stessa riformulazione - lo dico anche al Presidente della Commissione bilancio - facendo riferimento al comma 793 dell'articolo 1 della legge n. 197 del 2022, di fatto vi state riagganciando all'invarianza di spesa dell'intero provvedimento. Non c'è un euro, presidente Balboni, e se voi continuate a dire che questo è il tentativo di salvare la questione nazionale, ci costringete

che non c'è e vi chiederemo all'ultimo momento di approvarlo e di farlo passare. Il tema è uno solo: non c'è un centesimo. Da un lato Fratelli d'Italia vuole apparire il partito che salva la coesione e dall'altro c'è la Lega, che ha di fatto tradito la coesione e svenduto tutto per quell'obiettivo che è sotto gli occhi di tutti. Dobbiamo, insomma, assistere a un giochino tra i due principali partiti di maggioranza...

81 della Costituzione e poi nella stessa condizione trova una soluzione che in realtà una soluzione non è, sottoponete all'Assemblea il voto di alcuni principi, il che è come dire che il sole è bello e poi non ci dite come possiamo difenderci dalla pioggia. Il tema di fondo, Presidente, è che lei oggi con quella riformulazione ha consentito all'emendamento a prima

le relazioni da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, non è possibile non avere le relazioni tecniche, non è più sopportabile che diventi una sorta di valutazione orale. Noi abbiamo i rapporti

ha il mio sostegno totale, presidente Balboni, ma capisce che il tema è così grave che non può essere tirato fuori in Aula alla vigilia dell'approvazione di un provvedimento che è stato tutto condizionato dall'utilizzo del richiamo

modo tale da assumerci la responsabilità politica e di capire chi sta da una parte e chi sta dall'altra, ma quello che lei ha denunciato è quello che noi denunciamo dall'inizio della discussione che si è svolta su questo provvedimento. Per queste ragioni, Presidente, continuiamo a chiedere alla maggioranza di fermarsi.

Se mi è consentito di continuare... *(Commenti)*. Stiamo rispettando gli accordi, presidente Romeo.

Non abbiamo depositato testi, non abbiamo fatto nulla, quindi non capisco perché, dopo uno scontro istituzionale tra due Presidenti di Commissione, che nessuno dell'opposizione ha richiesto, dovremmo starcene in silenzio. Bastava che non ci fosse questo doppio intervento dei Presidenti e gli ultimi venticinque minuti di Aula non ci sarebbero stati. sarebbero stati. Ora, il Presidente della 1a Commissione, appartenente alla stessa forza politica del Presidente della 5a Commissione, le due Commissioni probabilmente più importanti nell'analisi della fase emendativa, dicono, caro Presidente della 5a, non puoi andare avanti così; e il secondo risponde: sì, Presidente della 1a, devo andare avanti così per questioni regolamentari. Credo che si debba porre rimedio a tutto questo. Ciò detto, e concludo, mi sento altresì di difendere l'operato del presidente Calandrini, che in tutti i passaggi ha sempre operato con grande rispetto per le opposizioni e per tutti i Gruppi politici che compongono la Commissione bilancio

e per riprendere quanto detto ora dal collega Patuanelli: è vero, c'è un'intesa tra le forze politiche di fare oggi il voto sugli emendamenti e martedì le dichiarazioni di voto. Io francamente però ritengo del tutto compatibile con l'*iter* che abbiamo immaginato, il fatto che si debba, alla luce di una novità vera che c'è stata stamattina in quest'Aula, cioè due interventi autorevolissimi del Presidente della 1a Commissione e del Presidente della 5a, entrambi evidentemente appartenenti alla maggioranza di Governo, avere un momento per approfondire questa cosa. Poi se preferite che la seduta della

non potete immaginare che sia semplicemente un problema dell'opposizione. È un problema di regole democratiche, di tenuta stessa del dibattito parlamentare. Io penso che sia un atto dovuto in sede di Giunta per il Regolamento affrontare la questione così come si è mostrata e in qualche modo porre un punto fermo a quello che francamente è un indirizzo che mette in una condizione di umiliazione tutti noi. Aggiungo una seconda rapidissima considerazione nel merito e mi

c'erano una serie di emendamenti, anche dell'opposizione, simili a questo, però, Presidente, davvero anche per quei pochi che stanno ascoltando - pochi o molti che siano, speriamo moltissimi

Ma immaginare che questo emendamento abbia significativamente cambiato il senso di questa proposta, francamente, presidente Balboni, questo no. Capisco la sua sofferenza, capisco la sofferenza del suo partito, che si chiama Fratelli d'Italia e e non Fratelli di mezza Italia *(Applausi)*, però capisce bene che c'è un limite a tutto. Per cui capisco la propaganda politica, capisco che dovete parlare al vostro elettorato, ma purtroppo questi emendamenti di cui stiamo discutendo non cambiano il tema di fondo di questa proposta di legge, che spacca profondamente il nostro Paese. Purtroppo, Presidente, il tema sull'invarianza di bilancio lo potete raccontare come volete, ma non risolve il problema che stiamo ponendo dall'inizio: se volete fare l'autonomia differenziata avreste dovuto dirci dal primo momento dove prendete i soldi per farla *(Applausi)*, innanzitutto per le Regioni del Sud e per colmare quei divari territoriali giganteschi, purtroppo, che invece inevitabilmente accentuerete.

delle cui modalità stiamo parlando non vengono definite sulla base del disegno di legge in esame, ma sono rimandate, secondo l'articolo 4 che abbiamo appena votato, a delle intese molteplici di atti bilaterali, tanti quanti saranno le Regioni che lo chiederanno. Questo rischia di creare davvero uno Stato che come potremmo definire Arlecchino, quando invece ci sarebbe bisogno di un quadro di coesione nazionale. Invito i colleghi a riflettere su questo

come poi vedremo anche all'articolo 8, di non rendere unitario questo processo. Sarebbe almeno importante che su tale

parere è contrario su tutti gli emendamenti. Sull'ordine del giorno G10.200, ci rimettiamo al Governo.

all'articolo 120 della Costituzione, al fine di garantire un sistema di continuità territoriale tra le Regioni della Sardegna e della Sicilia e il resto del Paese, adeguato ed efficace.

prima della votazione dell'articolo 10, che su questo articolo sono stati presentati alcuni degli emendamenti, poi diventati oggetto del dibattito della giornata di oggi e anche del confronto che prima c'è stato, aperto dal presidente Balboni, che sono stati dichiarati inammissibili. Lo dico, Presidente - poi il tema lo affronteremo perché c'era sostanza, soprattutto nell'emendamento 10.212 e lo dico soprattutto ai colleghi della maggioranza. Un Fondo di perequazione collegato all'autonomia era stato istituito con la legge di bilancio del 2021 il 30 dicembre del 2020 e il ministro Calderoli lo sa. Quel Fondo di perequazione era un atto di chiarezza e di trasparenza che al tempo del Governo Conte II era stato posto sul tavolo della Conferenza Stato-Regioni e della Conferenza unificata ed era la riprova che lo Stato faceva sul serio: metteva prima le risorse, poi definiva i tempi per la definizione dei livelli delle prestazioni e poi avrebbe seguito, autorizzato e accompagnato le intese con l'ultima parola del Parlamento. Signor Presidente, lo dico perché quel Fondo è stato cancellato con i tagli lineari dell'ultima legge di bilancio, quei 4,6 miliardi non ci sono più e ci ritroviamo una scatola vuota, che state portando all'approvazione con il voto finale che ci auguriamo avvenga il più tardi possibile, senza un solo centesimo che ci consenta di perequare le infrastrutture lo dico anche ai colleghi autonomisti - non solo per il Mezzogiorno, non solo per le aree interne, non solo per le aree di montagna, ma anche per le Regioni a Statuto speciale che rientravano in quella perequazione. Le Regioni a Statuto speciale non avranno nemmeno un centesimo con questo impianto e ovviamente non ci saranno risorse perché tutto questo provvedimento è a invarianza di spesa state portando avanti una riforma che, nella migliore delle ipotesi, dividerà il Paese e nella peggiore lo spaccherà definitivamente.

a quello che diceva il presidente Boccia, che non solo non c'è un euro in questo provvedimento, ma nella legge di bilancio quel Fondo perequativo è stato tagliato per tre miliardi e mezzo fino al 2033. *(Applausi)*. Quindi, non solo servirebbero 100 miliardi di euro per garantire e assicurare i LEP, ma è stato tagliato il Fondo perequativo, sono stati spostati 2,3 miliardi dal Fondo di sviluppo e coesione alla costruzione del Ponte sullo Stretto, sono stati persi 16 miliardi di euro dei progetti PNRR, di cui otto miliardi di progetti per il Sud,

degli atti di iniziativa delle Regioni già presentati al Governo, di cui sia stato avviato il confronto congiunto tra il Governo e la Regione interessata

vorrei avere un chiarimento è se la riformulazione che è stata proposta resuscita, ossia far tornare in vita delle intese stipulate da quattro Governi precedenti e da Consigli regionali e Presidenti di Regioni che oramai non hanno più alcuna legittimazione, oppure se è soltanto una garanzia di applicazione della vigente legge.

Non credo ce ne sia bisogno, Presidente. PRESIDENTE. Bene. Quindi, l'italiano è semplice: esamina senza alcuna preclusione in un modo o nell'altro. Lo esamina liberamente: vuol dire questo. L'interpretazione autentica

Allegato B)*. Come già comunicato, le dichiarazioni di voto finale avranno luogo nella seduta di martedì prossimo, alle ore 16,30, con la ripresa televisiva diretta.

la Presidente del Consiglio dei ministri ha detto ad Atreju, in un importante discorso che abbiamo seguito con attenzione,

La verità, però, il dato di fatto è che la rivendicazione orgogliosa della Presidente del Consiglio non può che vedere tutti noi felici. Noi siamo patrioti. Se l'Italia vince, non importa che il Governo sia di destra o di sinistra, facciamo festa tutti.

Expo 2030 l'Italia è arrivata terza su tre; non era facile e soprattutto non era mai successo: su 182 voti disponibili, ne abbiamo presi 17. Signor Ministro, io alla Farnesina una roba del genere non me la ricordo.

che andrà a Francoforte e non a Milano. Sul Tribunale unificato europeo dei brevetti ella ha espresso parole di grande entusiasmo, perché comunque una parte di quelle competenze andranno a Milano, ma l'articolo 87 dell'accordo istitutivo prevedeva che fossero tutte a Milano e che non fossero tolte, ad esempio, le competenze in materia di chimica e di metallurgia, Dio solo sa quanto questo sia importante per noi. Inoltre, signor Vice Presidente del Consiglio e Ministro degli affari esteri, per la Banca europea degli investimenti c'erano tre candidati: la spagnola, la danese e l'italiano. Come nelle barzellette, ma non fa ridere, siamo arrivati terzi: ha vinto Nadia Calviño. Signor Ministro degli affari esteri, io non vedo un'Italia che vince. L'unica vittoria l'ho vista in Coppa Davis, ma stento ad assegnarla alla vostra organizzazione, magari è meglio Sinner di lei su questo. su cosa sta vincendo l'Italia? Glielo chiedo perché noi, se l'Italia vince, siamo dalla vostra parte, perché noi siamo patrioti. Ho l'impressione che questo Governo vinca solo a parole. È in grado di smentirmi? Ne sarei felice.

capisco che siamo in campagna elettorale, ma purtroppo gli interroganti hanno commesso una leggerezza, perché i fatti sono molto diversi da quelli che vengono illustrati in Nell'ultimo anno il Governo ha rafforzato la posizione dell'Italia con una forte presenza nelle organizzazioni internazionali. senatore Renzi è impegnato in tante missioni internazionali, non segue le vicende e forse è rimasto a qualcosa di passato. In un quadro di elezioni competitive e di forte polarizzazione, il nostro è stato il Paese più votato negli organismi direttivi di numerose agenzie, a cominciare da quelle delle Nazioni Unite in settori per noi strategici. Lo stesso vale per gli incarichi apicali. Ricordo, ad esempio, signor Presidente, la nomina dell'ammiraglio Cavo Dragone a presidente del Comitato militare della NATO. Credo sia un incarico di grande rilievo per il nostro Paese all'interno dell'Alleanza

subito prima di diventare Ministro dell'economia e delle finanze dei Governi guidati dal senatore Renzi e dall'onorevole Gentiloni. Abbiamo anche assicurato la nomina di Maurizio Martina, anche lui ex Ministro del Governo del senatore Renzi, a vicedirettore generale della FAO.

È stato il nostro Governo - come ha ricordato il senatore Renzi - a portare a casa l'assegnazione a Milano di una sezione della divisione centrale del Tribunale unificato europeo dei brevetti e di competenze cruciali per il nostro tessuto industriale. risultato tutt'altro che scontato, perché il Tribunale avrebbe potuto avere solo due sedi, Parigi e Monaco di Baviera. Mi spiace dovermi ripetere anche sul caso della Libia: Tripoli aveva manifestato un'iniziale contrarietà, peraltro subito rientrata, all'ambasciatore dell'Unione europea, non a quello dell'Italia. C'è una differenza tra Unione europea e Italia, tra servizio esterno e ambasciatore d'Italia, che invece ha ottenuto l'immediato gradimento. Il voto su Expo 2030 ha confermato la potenza dei mezzi a disposizione di Riad, che il senatore Renzi ben conosce per i proficui rapporti che ha con l'Arabia Saudita e per la perfetta conoscenza della rivoluzione condotta dal sistema dell'Arabia Saudita. Io mi sarei aspettato un suo impegno per portare a casa magari il ritiro della candidatura saudita, grazie alle sue conoscenze, grazie alla sua amicizia, grazie ai proficui (forse per lui, ma non per l'Italia). Era una candidatura, quella, ereditata da altri e partita tardi, quando molti Paesi avevano già preso impegni con i nostri concorrenti. Abbiamo comunque dato tutti il massimo: il Capo dello Stato, il Governo, il Comune di Roma, la Regione e tanti altri. Ma era una missione impossibile; l'ha sottolineato lo stesso senatore Renzi, ricordando che l'ex sindaca di Roma (da lui definita "Dracula alla guida dell'AVIS") l'aveva lanciata a pochi anni da Expo Milano, per compensare la sua infelice rinuncia alle Olimpiadi. Comunque è chiaro che nelle candidature internazionali non si può sempre vincere. Il senatore Renzi ricorderà, ad esempio, la mancata assegnazione a Milano dell'Agenzia europea dei medicinali, nel 2017. Se forse, in quel famoso incontro al largo di Ventotene, fosse stato invitato anche il Primo Ministro spagnolo, forse la Spagna, invece di votare per l'Olanda, avrebbe votato per l'Italia. Quindi, a causa di un errore del Governo guidato dall'onorevole Renzi, abbiamo perso una agenzia fondamentale. A lui, esperto di gufi, diciamo: chi fa il tifo contro l'Italia per lucrare qualche consenso elettorale resterà deluso. In un anno il nostro Governo ha ridato all'Italia la centralità che merita e continuerà a battersi per difendere, non a parole, gli interessi nazionali. Signora Presidente, la ringrazio. Signor Ministro, fatico a trovare le parole - persino io, che di solito ho una certa facilità oratoria - per esprimere il mio imbarazzo Noi abbiamo presentato un'interrogazione partendo da un dato di fatto: a fronte di una frase della Presidente del Consiglio, negli ultimi due mesi abbiamo perso. Lei dice che non si può sempre vincere nelle competizioni internazionali. Ha ragione. Ma non si può nemmeno sempre perdere, come sta accadendo con lei. Signor Ministro, io sono il Ministro degli affari esteri? Perdo con diciassette voti l'Expo? Certo, posso venire in Aula e fare polemica contro l'opposizione. Ma forse convoco una riunione e capisco come si gestiscono meglio certi passaggi. Vede, signor Ministro, quando noi ci siamo trovati in una situazione difficile io ero *Premier* e al suo posto c'era Paolo Gentiloni - non eravamo sicuri di vincere contro l'Olanda per il seggio al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Cosa abbiamo fatto? Ci siamo fatti due conti e abbiamo fatto un accordo con Mark Rutte, per fare un anno per uno. Quando abbiamo portato a casa i risultati, questi non sono la Vice Segreteria dell'OCSE, che ci tocca tutte le volte; è una cosa - come lei giustamente ricordava - che non è nemmeno la vice direzione generale per Maurizio Martina. Per gli incarichi, quelli veri, signor Ministro, si fa squadra con le opposizioni. Lei è venuto qui e ha detto: capisco che siamo in campagna elettorale. Ce ne siamo accorti che lei è in campagna elettorale; non a caso si è occupato di bob

la gentilezza istituzionale di far parlare l'opposizione, perché le può riuscire, nei suoi comunicati stampa, di far tacere gli altri. Caro ministro Tajani, noi abbiamo avuto per lei parole di grande appoggio e sostegno, quando abbiamo cominciato un anno e mezzo fa. Non abbiamo mai detto una menzogna, come ha fatto lei rispetto al mio Governo - non era il mio Governo nel 2017, ma lo scoprirà con il tempo - e non abbiamo mai fatto il tifo contro l'Italia. Lei è venuto in quest'Aula e, anziché dire "ragazzi, è andata male, lavoriamo insieme per il futuro", ha offeso le istituzioni e ha offeso l'opposizione. Inizi a lavorare e smetta di far campagna elettorale: glielo chiede il Paese.

l'onorevole Ministro e tutti i membri del Governo presenti in Aula. Premesso che l'Italia ha assunto il 1° gennaio 2024 la Presidenza del G7 e ha annunciato che avrà fra le sue priorità il rispetto dell'ordine internazionale, profondamente scosso dalla guerra russa in Ucraina e dal conflitto in Medio Oriente, dopo gli attacchi terroristici di Hamas del 7 ottobre, il terrorismo che ha colpito Israele, e l'inizio delle operazioni israeliane nella striscia di Gaza, i ribelli yemeniti di Ansar Allah, cosiddetti Houthi, hanno cominciato a condurre attacchi contro le navi in transito nel mar Rosso, in particolare nello stretto di Bab el-Mandeb, mettendo a rischio la libertà e la sicurezza della navigazione lungo una delle rotte commerciali più importanti al mondo e arrecando danno alle compagnie di navigazione, molte delle quali hanno deciso di sospendere le rotte attraverso il mar Rosso e il canale di Suez. La crisi sta spingendo le compagnie di navigazione a rinunciare all'ingresso nel Mediterraneo optando per i porti del Nord Europa. La crisi rischia così di ridurre l'importanza commerciale dei principali porti italiani: pensiamo a Trieste e a tutta la dorsale adriatica. Noi rischiamo, dunque, di vedere inficiata la centralità del Mediterraneo nella rotta commerciale che collega l'Asia all'Europa e agli Stati Uniti. Appaiono, inoltre, concreti i rischi di un'estensione del conflitto in Medio Oriente, riferimento allo Yemen, e il pericolo di vanificare i progressi compiuti negli ultimi mesi per la pacificazione intra-yemenita. Il 22 gennaio a Bruxelles si terrà la riunione del Consiglio affari esteri dell'Unione europea, al cui ordine del giorno è prevista la discussione sulla situazione nel mar Rosso. Alla luce di quanto esposto, che è del resto ben noto, con tutte le preoccupazioni che la comunità internazionale e anche gli italiani avvertono, chiediamo quali sono le iniziative che lei, signor Ministro, intende intraprendere per rafforzare la sicurezza nella regione e per preservare la libertà di navigazione e gli interessi economici italiani. di navigazione lungo una delle rotte commerciali più importanti del mondo. Danneggiano le nostre compagnie di navigazione e i porti italiani di Gioia Tauro, Brindisi, Taranto, Trieste. Genova, solo per citarne alcuni. Sul piano interno, stiamo lavorando con tutte le amministrazioni interessate. Per il Governo è una assoluta priorità assicurare l'ordinato svolgimento dei flussi commerciali e, allo stesso tempo, la sicurezza nella regione. A livello internazionale, stiamo seguendo attivamente tutti gli sviluppi insieme ai *partner*, in particolare, in ambito dell'Unione europea e G7. Vogliamo ripristinare la sicurezza della navigazione nell'area, evitare una pericolosa estensione del conflitto in Medio Oriente e salvaguardare i passi avanti degli ultimi mesi per la pace in Yemen tra il Governo riconosciuto e i ribelli Houthi. La risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 gennaio condanna fermamente gli attacchi Houthi e sottolinea il diritto degli Stati ad agire per la difesa del proprio naviglio, nel rispetto del diritto internazionale. Abbiamo assicurato il nostro sostegno politico alle operazioni angloamericane in Yemen, volte a fiaccare le capacità di attacco degli Houthi. Fin dall'inizio abbiamo accolto con favore l'annuncio statunitense dell'avvio della missione *Prosperity Guardian*, sostenuta da una coalizione politica di oltre quaranta Paesi, tra cui appunto l'Italia. Il Ministero della difesa ha messo a disposizione, con compiti di supporto associato, la fregata Virginio Fasan, che già da dicembre avevamo spostato nell'area delle operazioni e, più di recente, la fregata Federico Martinengo. Il Governo italiano non partecipa agli attacchi anglo americani contro gli ma promuove una risposta europea che possa tutelare le nostre navi mercantili. È importante essere tempestivi e, allo stesso tempo, assicurare il coordinamento tra le diverse operazioni nella regione e un raccordo con i Paesi che su quei mari si affacciano e condividono il nostro interesse alla sicurezza e alla stabilità. Ne ho parlato ieri con il ministro degli affari esteri giordano Safadi e ne parlerò con l'omologo egiziano Shoukry. Egitto e Giordania sono, infatti, i due Paesi della regione più direttamente colpiti dalla crisi del mar Rosso. Per concludere, l'azione diplomatica deve andare avanti di pari passo con quella militare. Rimane fondamentale mantenere canali di dialogo aperti con tutti gli attori che possono esercitare la propria influenza nella regione. Sullo sfondo, resta la guerra a Gaza. Vogliamo evitare ulteriori *escalation* in Medio Oriente. Le recenti tensioni tra Iran, Iraq, Siria e Pakistan sono un segnale preoccupante. Nei prossimi giorni sarò a Bruxelles per discutere questi temi con i *partner* europei e poi in Libano, Israele e Palestina, per portare un messaggio di pace e di dialogo.

recentemente, in occasione di dibattiti pubblici, incontri di categorie ed eventi mediatici, di riscontrare come gli armatori italiani abbiano riconosciuto l'impegno della Marina italiana che sta dando tutta l'assistenza necessaria in una fase molto difficile, con l'equilibrio che lei anche oggi ha ricordato che l'Italia ha tenuto in tutto questo quadrante, sia evitando aggressioni preventive, sia essendo pronta a qualsiasi reazione a tutela delle nostre navi e dei commerci, che sono molto importanti per la proiezione mediterranea e per i porti, come ricordavo prima, da Trieste in giù, che rischiano di essere sacrificati rispetto ad altre rotte del Nord Europa raggiungibili circumnavigando l'Africa. È lo stesso equilibrio che lei ha dimostrato anche nella vicenda di Gaza ed Israele, con una posizione chiarissima a sostegno del popolo e dello Stato di Israele aggredito, ma anche attento a far sì che, nella dinamica tragica di quell'area,

C'è chi gira il mondo per la propria attività - per carità, rispettabilissima - e c'è chi gira il mondo per rappresentare gli interessi dell'Italia, gli interessi della pace e anche la nostra autorevolezza che, come prima ricordato, si farà sentire anche nel vertice della NATO nei prossimi mesi,

ma l'Italia sa farsi ascoltare e rispettare. So che anche nei prossimi giorni la attende un intenso programma che sarà utile per far sì che il mondo ragioni. Continui quindi a viaggiare per le nobili ragioni. Gli altri viaggiano per altre esigenze.

Signor Ministro, come è stato detto pocanzi, è ormai evidente che l'*escalation* del conflitto israelo-palestinese si ripercuote in maniera importante nelle dinamiche geopolitiche del quadrante meridionale. In particolare, poi, come è già stato detto, l'aumento delle azioni militari della milizia yemenita degli Houthi, sostenuta tra l'altro - questo dobbiamo sottolinearlo - dall'Iran, vede questi ripetuti attacchi, in particolare nei confronti della navigazione commerciale nell'area del mar Rosso. Nonostante una pronta azione anche militare condotta dagli Stati Uniti, ma anche dalla Gran Bretagna, che è volta evidentemente a diminuire questi atti, questi atti, soprattutto con iniziative militari davvero importanti, che hanno indebolito anche le forze degli Houthi, le compagnie di navigazione hanno ormai deciso di circumnavigare l'Africa e quindi le conseguenze le conseguenze sono inevitabili: non solo l'aumento dei costi, che evidentemente hanno ripercussioni importanti su tutte le nostre imprese, ma anche poi l'abbandono dell'area del Mediterraneo da parte di questa navigazione.

quali siano le interlocuzioni che sono state avviate con gli alleati internazionali e con tutti i Paesi europei al fine di attuare delle iniziative concrete per mettere in sicurezza quest'area,

La minaccia Houthi sta già determinando una diminuzione delle navi che transitano per il mar Rosso, passate da 400 a 250 al giorno. Sono aumentati, e non di poco, i costi assicurativi e si allungano i tempi di percorrenza. come ha sottolineato anche l'interrogante, della competitività dei nostri porti, e c'è il rischio anche di un aumento dei prezzi per il consumatore finale. Il Governo intende agire in modo rapido e pragmatico. Stiamo già promuovendo una risposta europea alla crisi nel mar Rosso. Vogliamo rafforzare la presenza militare europea nell'area per tutelare la libertà di navigazione e dei traffici. Dobbiamo partire dall'esperienza maturata nelle operazioni esistenti per pianificare una nuova missione europea. Le missioni ora schierate nella regione sono due. Una è Atalanta, creata nel 2008 dall'Unione europea, che ha il compito principale di difesa dalla pirateria in un'area che va dal mar Rosso al Corno d'Africa. Emasoh-Agenor, è quella che presidia lo Stretto di Hormuz, punto di accesso nel Golfo Persico, lanciata nel 2020 da una coalizione di nove Paesi europei, Italia inclusa. Lunedì parteciperò a Bruxelles al Consiglio affari esteri. Ho parlato con la ministra degli affari esteri tedesca Baerbock e con il nuovo ministro francese Séjourné. Con Parigi e Berlino stiamo portando avanti un'iniziativa congiunta: far leva su assetti già presenti nell'area permette una risposta più rapida. Il rafforzamento della missione Atalanta vede però la contrarietà della Spagna che ne ospita il quartier generale. Stiamo quindi lavorando, signora Presidente, a una nuova missione, Aspis, che ingloberà Emasoh-Agenor, già operativa nello Stretto di Hormuz, e opererà anche nel mar Rosso e Golfo di Aden. Potrebbero partecipare a questa nuova missione anche i Paesi non membri dell'Unione europea. Il nostro obiettivo è quello di prendere una decisione politica già lunedì, in modo che la missione possa essere operativa al più presto. Sarà una missione non di attacco, ma di difesa. Le navi militari europee interverrebbero a tutela dei mercantili cui fanno la scorta. L'operazione punta a creare un meccanismo di dissuasione per difendere il traffico marittimo in tutta l'area fino a Suez. Più in generale, la situazione in corso ripropone l'esigenza per l'Unione europea di fare passi avanti nell'ambito della difesa per rafforzare il ruolo di fornitore di sicurezza globale. signor Ministro, ancora una volta lei è stato assolutamente esaustivo. Come ha confermato ritengo che la sicurezza del mar Rosso è fondamentale, evidentemente per l'interesse nazionale, l'interesse del nostro Paese. Ci tengo poi a sottolineare e a ribadire con forza che è importantissimo che continuiamo a tenere alta la bandiera del Paese anche nella difesa degli interessi nazionali, in Italia ma soprattutto all'estero, e quindi anche nell'area allargata

attivi ed efficaci per dimostrare che il nostro Paese è protagonista, a differenza di quanto altri dicono, ed ha riconquistato un ruolo importante a livello internazionale. Possiamo fare di più e meglio? Certamente sì, però siamo sulla buona strada. In questo noi vi incoraggiamo e vi siamo vicini. Vorrei poi sottolineare che questa mia sensibilità, questa nostra sensibilità è dettata, come lei ha detto, anche dal fatto - mi riferisco al mar Rosso e ai traffici - che evidentemente i nostri porti sono particolarmente esposti. Io vengo dal Friuli Venezia Giulia. Il porto di Trieste oggi è probabilmente il primo porto in Italia per traffici che arrivano anche da quei territori, quindi l'attenzione che dobbiamo porre, anche rispetto alla *devolution* in questo senso, ai territori e al PIL locale è assolutamente importante. La difesa dell'interesse nazionale

Dal punto di vista economico si sono già manifestate le conseguenze sui noli marittimi del trasporto *container*, con un aumento settimanale in alcuni casi addirittura decuplicato. Molta preoccupazione è stata dichiarata da parte del presidente dell'ABI, Antonio Patuelli, per i traffici delle merci delle merci nel Mediterraneo. Le principali compagnie di navigazione dichiarano di evitare il mar Rosso e il Canale di Suez per ragioni di sicurezza, dando adito anche a fenomeni speculativi, con impennate significative rispetto alla rilevazione del 21 dicembre del 2023. Zeno D'Agostino, presidente del porto di Trieste, ha segnalato che, se la situazione dovesse protrarsi, il rischio è che le navi, una volta circumnavigata l'Africa, puntino direttamente sui porti del Nord Europa a discapito del Mediterraneo e le stesse preoccupazioni affliggono Genova e gli altri porti italiani. Un perdurante, massiccio massiccio blocco della libera navigazione sulla rotta di Suez costituirebbe un attacco alla sicurezza dell'Unione europea e danneggerebbe in modo pesantissimo il nostro Paese e gli altri Paesi del Mediterraneo. L'Italia è presente nell'area con due unità navali. Il Governo italiano ha precisato di non aver partecipato partecipato agli attacchi condotti da Stati Uniti e Gran Bretagna, perché - cito - «non possiamo mettere in atto azioni di guerra senza un dibattito in Parlamento». Tra le operazioni già esistenti nell'area figura una missione navale europea, cui partecipa anche l'Italia al largo della Somalia, con l'obiettivo di contrastare attività di pirateria. Da diverse settimane l'Unione europea sta studiando la possibilità di avviare una missione militare navale a protezione delle navi commerciali in mar Rosso. Il Ministro degli affari esteri ha reso noto che il Governo si sta adoperando perché possa esserci una missione militare europea per proteggere i traffici commerciali. Si chiede quindi di sapere se il Ministro non ritenga opportuno attivarsi tempestivamente al fine di definire una strategia finalizzata a ottimizzare, nel brevissimo termine, l'impiego delle unità navali e di altri strumenti dissuasivi a protezione dei traffici; quale sia la situazione attuale e in prospettiva delle Autorità di sistema portuale maggiormente colpite. Si chiede altresì di aprire subito un'interlocuzione anche con i soggetti pubblici e privati coinvolti nelle filiere del trasporto, della logistica e dello *shipping*. Si chiede valuti improrogabile, come appena detto da lei, alla luce della situazione internazionale, l'assunzione di una risoluzione a livello di Unione europea per procedere all'integrazione europea dell'energia e della politica estera, nonché a un accordo sullo strumento militare europeo, sul suo finanziamento e sul

come ho già sottolineato, la riduzione del traffico marittimo nel mar Rosso a causa degli attacchi degli Houthi ci preoccupa. Per Suez transita circa il 40 per cento del nostro interscambio commerciale marittimo. Nelle scorse settimane è aumentato sensibilmente il rischio di navigazione in quell'area, in particolare dello Stretto di Bab el-Mandeb, per gli attacchi condotti con missili e droni ai danni delle navi commerciali in transito. Gli attacchi stanno mettendo a rischio una delle rotte commerciali più importanti al mondo, soprattutto per quanto riguarda i rifornimenti energetici dell'Europa meridionale, Italia inclusa, provenienti dai Paesi del Golfo. Nel complesso gli attacchi sono stati circa 30, l'ultimo dei quali l'altro ieri, contro la nave di proprietà dell'armatore greco, battente bandiera maltese. Come conseguenza, i flussi commerciali sono stati riorientati. Il volume degli scambi attraverso Suez è diminuito del 28 per cento su base annua fra l'ultima settimana di dicembre e la prima settimana di gennaio; i volumi degli scambi attraverso il Capo di Buona Speranza sono invece aumentati del 67 Fare il periplo dell'Africa significa un aumento anche di quindici giorni dei tempi di consegna. Ciò comporta un aumento dei costi della logistica e quindi dei prezzi delle merci e rischia di penalizzare fortemente i nostri porti. Siamo in contatto, come ho detto, con i vertici delle principali associazioni di categoria del settore, armatori e porti. C'è preoccupazione che l'attuale situazione di crisi possa, ahimè, protrarsi. Non dimentichiamo il settore delle crociere fiorenti in quell'area. I problemi di sicurezza nel mar Rosso hanno un impatto e gli operatori temono una perdita di fatturato. Il Governo sta lavorando per tutelare i nostri interessi economici ed evitare interruzioni delle rotte di approvvigionamento di materie prime, semilavorati e prodotti finiti. Confermo che il Governo sta promuovendo una risposta europea alla crisi del mar Rosso. Come ho detto precedentemente in quest'Aula, la nostra proposta è quella di allargare le competenze della missione militare che protegge la navigazione nello Stretto di Hormuz per arrivare fino a Suez. Questo per guadagnare tempo e non dover ridar vita a una nuova missione militare, che richiederebbe invece tempi più lunghi. La situazione in corso ripropone l'esigenza per l'Unione europea di fare passi avanti nell'ambito della difesa europea. Ho dedicato parte della mia vita a battermi per questo e, quindi, sono assolutamente d'accordo. Non si può avere una politica estera europea se non c'è la difesa europea. Vogliamo un'Europa che abbia un rapporto paritario con gli Stati Uniti e con la NATO e vogliamo un deciso rafforzamento della cooperazione tra Unione europea e NATO, sempre più essenziale nell'attuale contesto internazionale. Bisogna individuare progetti di interesse comune e favorire economie di scala. Dobbiamo porre fine a duplicazioni e incompatibilità. L'obiettivo finale è quello di un esercito europeo capace di condurre missioni di pace e intervenire in tempi molto rapidi.

quella che ha seguito il grido d'allarme degli operatori del settore. È chiaro che l'attacco degli Houti è destabilizzante Houti è destabilizzante sotto il profilo non solo della sicurezza ma - come ha detto la collega - anche economico, perché non solo i traffici marittimi ne vengono vulnerati e le compagnie marittime sono obbligate sostanzialmente a circumnavigare l'Africa, ma anche la portualità italiana ne esce con gravissimi danni. Dunque, la strada è quella che abbiamo indicato assieme; l'ha ricordata la collega e lei ha la stessa cosa: la strada è quella europea. Non possiamo pensare a individualità che non avrebbero senso, né possiamo pensare a bellicismi che sarebbero fuori dal seminato. Dobbiamo lavorare perché una missione europea garantisca i traffici commerciali.

Credo - e il Gruppo che rappresento in questo *question time* ne è convinto - che non ci può essere un'Europa credibile se al polmone economico non segue e non si affianca un'anima, che è la politica estera e di difesa. La politica estera e di difesa sono giustamente connesse perché non c'è politica estera efficace se non c'è un'integrazione con il sistema di difesa. Chiunque vinca le elezioni americane - lo vediamo sullo sfondo ed è inutile che ci facciamo tanti interrogativi su chi vincerà, perché lo vedremo - e in ogni caso dietro lo *slogan* "America First" c'è una richiesta dell'opinione pubblica americana affinché la stessa Europa esca da uno stato di infantilismo politico e si assuma le sue responsabilità. Noi siamo pronti a fare questo. Bisogna che l'Italia, tutto il sistema Italia, maggioranza e opposizione, lavori perché le prossime elezioni europee siano una spinta nella direzione della difesa comune europea. D'altronde, certi momenti drammatici drammatici consentono agli uomini di dare il meglio delle proprie individualità. Mi auguro pertanto che anche questa vicenda costituisca una spinta perché noi europei veramente usciamo dall'infantilismo e dalla minore età per diventare adulti. Termino

russi e turchi. Sia gli italiani che i francesi e collegialmente tutti gli europei hanno una posizione irrilevante. La colpa è certamente non di questo Governo, ma di un insieme del nostro passato che ci portiamo dietro, e oggi dobbiamo assieme fare passi avanti.

Tra le varie misure introdotte in questi anni vi è il cosiddetto Daspo urbano, volto a vietare l'accesso dei soggetti autori di condotte lesive in specifiche aree pubbliche. Con il cosiddetto decreto Caivano il Daspo urbano è stato esteso anche nei confronti di soggetti che abbiano compiuto quattordici anni. In caso di inottemperanza del divieto, il contravventore è punito con l'arresto da sei mesi a un anno. Tuttavia le città continuano a non essere sicure, specialmente in prossimità di particolari luoghi come le stazioni ferroviarie, le piazze, i parchi cittadini e i dintorni dei locali notturni. Da quel che risulta, gli strumenti a disposizione dei questori, tra cui il Daspo urbano, nei casi di reiterazione delle condotte sono ad oggi scarsamente utilizzati. altresì che come già segnalato all'interno di una precedente interrogazione, l'Alto Adige-Südtirol, al pari di altre realtà territoriali, è diventato ormai teatro di ripetuti episodi di violenza, commessi anche da minori minori e che interessano in particolare le città di Merano e Bolzano, dove lo spaccio di droga, risse e lesioni aggravate sono ormai all'ordine del giorno, giorno, si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo possa comunicare il numero dei provvedimenti di allontanamento e di "DASPO urbano" complessivamente adottati nell'ultimo anno, con riferimento sia all'intero territorio nazionale, sia all'Alto Adige-Südtirol e al Trentino, in particolare, alle città di Merano, Bolzano e Trento e se, in generale, sia a conoscenza dei motivi che ostano all'adozione, da parte degli organi incaricati, di tali provvedimenti.

una priorità per il Governo che sta dedicando a questo obiettivo un impegno straordinario ed ingenti risorse, come avrò modo di riferire anche in risposta alle altre interrogazioni della seduta odierna. Sul piano normativo abbiamo sin dall'inizio adottato misure specifiche, con particolari riferimento ai divieti di accesso in determinati luoghi e aeree urbane, a cui gli interroganti fanno riferimento; con il decreto Caivano ne abbiamo affinato l'operatività mediante l'ampliamento del raggio di applicazione della platea dei destinatari, anche inasprendo il regime sanzionatorio. Quanto ai dati richiesti, evidenzio che dalla banca dati CED interforze risultano adottati nel 2023 sul territorio nazionale complessivamente 11.083 provvedimenti di allontanamento. In Provincia di Trento sono stati tre i provvedimenti di allontanamento, tutti riferiti al Comune capoluogo. Invece, per quanto riguarda la Provincia di Bolzano, risultano 146 provvedimenti di allontanamento, di cui 143 relativi al Comune capoluogo, 2 al Comune di Brunico e 1 al Comune di Bressanone. In relazione poi ai provvedimenti di Daspo urbano e del divieto di accesso al locale di pubblici esercizi, nel 2023 il CED interforze registra complessivamente 2.902 provvedimenti; di essi 874 sono relativi al divieto di accesso a particolari luoghi, 441 sono riferibili al divieto di accesso a locali pubblici ai fini di prevenzione dello spaccio di stupefacenti, 1.532 alle disposizioni per la prevenzione di disordini negli esercizi pubblici e 500 risultano adottati in attuazione delle nuove disposizioni introdotte dal cosiddetto decreto Caivano. In particolare nella Provincia di Trento non risultano provvedimenti di Daspo urbano adottati dal questore, mentre in Provincia di Bolzano risultano adottati 18 Daspo urbano, di cui 12 relativi al Comune capoluogo, 3 al Comune di Merano, 2 al Comune di Corvara in Badia e 1 al Comune di Brunico. L'attenzione del Governo sui temi evidenziati resta alta, a partire dal controllo del territorio e dalle misure di prevenzione e contrasto di ogni forma di illegalità. Ricordo infine che ulteriori interventi normativi, sempre in materia di sicurezza urbana, sono stati previsti dal disegno di legge approvato dal Consiglio dei ministri dello scorso 16 novembre, e vanno tra l'altro nella direzione di estendere la possibilità di disporre il Daspo anche per vietare l'accesso alle aree di infrastrutture e pertinenza del trasporto pubblico ai soggetti denunciati o condannati per reati contro la persona o il patrimonio, le stazioni in particolare. *(Applausi)*. PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire in replica la senatrice Unterberger,

a quanti delinquono non succede niente: vengono fermati, ma il giorno dopo vengono visti di nuovo al posto dove hanno commesso il reato, dove hanno commesso le violenze.

della Provincia di Napoli si assiste quotidianamente a episodi di furto con scasso che stanno mettendo in ginocchio e piegando i commercianti dell'area, che non solo si vedono arrecare danni per migliaia di euro, ma assistono anche inermi all'impossibilità di avere garantite sicurezza e prevenzione. A Roma, signor Ministro, si sono registrati due omicidi in tre giorni: un quattordicenne è stato ucciso nel parcheggio della metro e un trentatreenne è stato freddato a colpi di pistola sotto casa. A questi due fatti si aggiunge quello di Anzio, ovvero il ferimento di un diciassettenne con un colpo di pistola mentre rientrava a casa da scuola. Vi è poi il caso di Michelle, signor Ministro, una bambina di sei anni morta folgorata in un campo rom in una cittadina a nord di Napoli, Giugliano; un campo rom che da troppo tempo attende di essere smantellato, perché è un luogo di degenerazione e di malaffare. Dopo la morte della piccola, parenti e amici della famiglia hanno assaltato l'ospedale e danneggiato anche l'auto della polizia. Sono atti di criminalità e di violenza efferata che lasciano sgomenti, ma che non possono cadere nell'indifferenza. A Mergellina, sempre Napoli, nel marzo 2023 Francesco Pio Maimone, un pizzaiolo napoletano di appena diciotto anni, fu ucciso nel mezzo di una rissa scatenata per futili motivi: qualcuno era stato calpestato e gli si era sporcata la scarpa. Non si può non ricordare l'omicidio di Giovanbattista Cutolo, il musicista dell'orchestra Scarlatti Young, di ventiquattro anni, ucciso a colpi di pistola nell'agosto del 2023 in Piazza Municipio a Napoli per il parcheggio di uno *scooter*. Si chiede di sapere, in considerazione dell'aumento degli episodi di criminalità, violenza e delinquenza che stanno interessando la città di Roma e la Provincia di Napoli, quali iniziative il Governo intende adottare per migliorare la sicurezza di queste realtà e dei loro cittadini, quali azioni concrete intenda adottare il Ministro in indirizzo per rafforzare la prevenzione della criminalità e migliorare la sicurezza delle città e dei cittadini; se e come si intende aumentare la presenza delle Forze dell'ordine nei quartieri più a rischio e quali risorse siano state messe a disposizione per rafforzare la presenza delle stesse sul territorio. Si chiede altresì quali siano le iniziative per garantire la sicurezza nelle zone a rischio delle città, quali periferie e quartieri più colpiti dalla criminalità organizzata.

le linee d'intervento attivate d'intesa con i sindaci sono finalizzate ad assicurare una sempre più capillare e visibile presenza delle Forze dell'ordine, anche mediante la realizzazione sistematica di operazioni interforze ad alto impatto che stanno producendo risultati a mio giudizio - positivi in termini di capacità di controllo del territorio e di prevenzione e contrasto di ogni forma di illegalità. Continueranno in tale direzione anche tutte le azioni già intraprese per contrastare il fenomeno delle occupazioni abusive di immobili, per smantellare le piazze di spaccio, per restituire alla piena fruibilità dei cittadini gli spazi urbani che presentano criticità legate a condizioni di degrado. Per dare dei numeri, dal 1° gennaio 2023 al 17 gennaio di quest'anno a Roma sono stati effettuati 140 servizi denominati ad alto impatto e a Napoli 135. Complessivamente sono stati impiegati 18.854 operatori delle Forze di polizia, 1.173 della Polizia locale, 2.167 unità di personale che hanno proceduto all'arresto di 639 persone e alla denuncia di 2.805 persone. Sono state altresì adottate 298 misure di prevenzione personale e 95 provvedimenti di espulsione dal territorio nazionale nei confronti di cittadini stranieri. Quanto agli episodi avvenuti nelle due città citate nell'interrogazione, l'azione investigativa sinora svolta ha consentito di individuare diversi soggetti coinvolti a vario titolo nelle azioni criminali, mentre sono tuttora in corso le indagini volte ad individuare i responsabili dell'omicidio avvenuto lo scorso 15 gennaio nel quartiere Corviale di Roma. Oggi a Roma domani a Napoli i prefetti hanno convocato i rispettivi comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza pubblica, proprio al fine di approfondire i recenti episodi citati dall'interrogante. Ne attendo gli esiti. L'azione di prevenzione e repressione e le attività info-investigative su un piano più generale devono essere affiancate - come dimostra l'impegno che si sta realizzando a Caivano e non solo - da quelle per la rigenerazione e la riqualificazione urbana, mediante il coinvolgimento sinergico dei vari livelli di governo del territorio, con il fine di spezzare l'intreccio tra degrado e illegalità e superare quei fenomeni di marginalità sociale in cui le criminalità A tali fini, oltre agli importanti investimenti derivanti dal PNRR, i Comuni potranno utilizzare, grazie al mio decreto del 22 dicembre scorso, ulteriori risorse provenienti dal fondo per la sicurezza urbana, di cui (riferite alla sola annualità del 2023) per Roma circa 6 milioni milioni e mezzo e per Napoli circa 4 milioni. Continua inoltre il potenziamento degli organici delle Forze di polizia, avviato con la legge di bilancio per il 2023 e continuato poi con l'ultima legge di bilancio. Con riferimento alla Polizia di Stato, a Roma, nel corrente mese, il personale è stato incrementato di 123 effettivi, dei quali 70 assegnati alla questura; mentre a Napoli il potenziamento è stato di 165 unità, delle quali 150 assegnate alla questura. Per l'Arma dei carabinieri, nel corso del 2023, il saldo tra assegnazioni effettuate e trasferimenti in altre Province registra a Roma un incremento di 321 unità e a Napoli di A ciò, da ultimo, si aggiungono i militari del contingente ordinario dell'operazione "Strade Sicure", che, per effetto di quanto stabilito con la legge di bilancio, per Roma verranno incrementati di 100 unità, giungendo a complessive 1.394 unità, mentre a Napoli l'incremento di ulteriori 45 unità porterà la forza disponibile a 658 unità.

deve mettere in moto un meccanismo tale da poter garantire ancora e maggiormente quelle risorse necessarie al controllo del territorio, perché è difficile. Ritengo sia cruciale adottare un approccio globale che affronti non solo le conseguenze della criminalità diffusa, ma anche le sue radici, compresi i fattori sociali, economici e culturali che favoriscono la sua diffusione. Solo attraverso uno sforzo coordinato e sostenuto sarà possibile poi affrontare in modo efficace l'emergenza criminalità. Mi consenta, signor Ministro, a proposito di tale problema, di dirle che la sicurezza dei cittadini non va solo garantita, ma va fatta anche percepire. Le posso assicurare che in questo momento non è facile vivere nei nostri territori, che sembrano quasi di di frontiera. Soprattutto mi corre l'obbligo di dire che di certo non ha aiutato, da parte del Governo, non mettere ancora in atto quelle politiche attive del lavoro

molti italiani sono preoccupati di poter subire furti, molestie o aggressioni, per la propria sicurezza, in particolare nei luoghi ad alta frequentazione, e tra questi, soprattutto, nelle stazioni ferroviarie. Il potenziamento della sicurezza in prossimità delle stazioni, dove si concentrano tradizionalmente degrado ed emarginazione e, conseguentemente, criminalità e violenza, risulta imprescindibile per garantire il diritto alla mobilità e la fruibilità degli spazi da parte della comunità, sia nelle grandi città sia nelle città più piccole. Si consideri che nelle arre di Roma Termini e Milano Centrale transitano ogni giorno circa un milione di viaggiatori,

di 800 unità preposte all'attività di controllo nelle stazioni ferroviarie, si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo abbia posto in essere o intenda intraprendere al fine di garantire adeguati livelli di sicurezza nelle aree ferroviarie italiane, in particolare in quelle in cui si concentra il maggior transito di passeggeri.

ad alta frequentazione di pubblico, come le stazioni ferroviarie, svolge una importante funzione di deterrenza dell'illegalità. Per questo abbiamo attivato da subito operazioni interforze ad alto impatto - le abbiamo definite così - che vedono l'impiego di personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza, nonché della Polizia locale e il supporto di tutti gli altri attori interessati, diretti prioritariamente al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, dell'abusivismo commerciale, nonché al controllo della permanenza regolare degli stranieri sul territorio nazionale. Dal 16 gennaio 2023 al 16 gennaio di quest'anno, il personale delle Forze di polizia impiegato nei servizi è stato di 33.590 unità, cui si sono aggiunti 2.257 appartenenti alla Polizia municipale e 2.079 dipendenti di altri enti, quali ASL, ispettorati del lavoro e aziende municipalizzate: questo solo per gli ambiti ferroviari. Su un totale di 382.350 persone controllate, di cui 151.419 straniere, 670 sono state arrestate e 3.919 denunciate; tra queste, 1.835 per violazioni di natura amministrativa. I controlli hanno riguardato anche 38.096 veicoli e 6.722 esercizi pubblici, dove sono stati individuati 582 lavoratori in nero e irregolari. Gli stranieri espulsi sono stati 822, dei quali 88 accompagnati presso i CPR e 8 direttamente alla frontiera. All'esito delle attività di polizia sono state disposte 515 misure di prevenzione personale ed accertate 5.332 violazioni, di cui oltre 2.230 di natura fiscale. Inoltre, sono stati sequestrati denaro, merce contraffatta o insicura, stupefacenti, veicoli e armi. Questo per dare il il panorama dei risultati dell'impegno profuso. Quindi, l'azione delle Forze di polizia sta restituendo risultati positivi in termini di riduzione dei reati che maggiormente si consumano nei predetti contesti urbani. Va però sottolineato che, anche quando le attività di prevenzione non sono riuscite ad impedirne la commissione, la presenza rafforzata delle Forze di polizia ha reso comunque possibile assicurare tempestivamente alla giustizia i responsabili di fatti gravi. Al fine di intensificare ulteriormente la cornice di sicurezza, con l'ultima legge di bilancio abbiamo rafforzato la presenza dei militari nelle stazioni, finanziando un'aliquota di personale dedicato di 800 unità, di cui beneficeranno in gran parte, ovviamente, le stazioni di Roma e Milano. Abbiamo, altresì, incrementato il contingente dei militari dell'operazione "Strade Sicure", che raggiungerà le 6.000 unità rispetto alle 5.000 originariamente previste lungo questa linea tracciata. A breve incontrerò i sindaci delle tre maggiori aree metropolitane, per estendere le operazioni straordinarie di controllo del territorio, che hanno portato a questi risultati e numeri, anche alle aree limitrofe alle stazioni, allo scopo di introdurre più incisive misure di prevenzione, complementari al piano coordinato di controllo del territorio in quelle città ed in grado di aumentare la percezione di sicurezza dei cittadini, soprattutto negli orari più a rischio.

dichiaro assolutamente soddisfatto della sua risposta. Siamo molto contenti del lavoro che sta svolgendo il Governo e, in particolare, il il Ministero che lei così autorevolmente guida. È chiaro che in pochi mesi o in pochi anni è impossibile risolvere un problema così grave come quello della sicurezza nei luoghi pubblici che purtroppo, colpevolmente, è stato così a lungo trascurato nel recente e anche nel meno recente passato. Il Gruppo Fratelli d'Italia è al fianco del Governo per tutte le iniziative che vorrà intraprendere per garantire la sicurezza ai cittadini. Tutti sappiamo che senza sicurezza non c'è nemmeno libertà e, se non si garantiscono le condizioni minime di civile convivenza ai cittadini, nessuno si sentirà davvero libero. La ringraziamo, quindi, per il lavoro che

Signor Presidente, onorevoli colleghi, da abruzzese e da rappresentante delle istituzioni, oggi non posso non ricordare che il 18 gennaio segna una ferita indelebile nella storia della nostra amata terra d'Abruzzo. Sette anni fa, a Farindola, un piccolo Comune ai piedi del Gran Sasso, si consumava una terribile tragedia, la tragedia di Rigopiano. In quella giornata la natura sembrava essersi accanita su tutto l'Abruzzo e in quell'angolo bellissimo della nostra terra si verificavano una bufera di neve senza precedenti, con accumuli che in alcuni punti superavano i tre metri di altezza e, come se non bastasse, anche scosse di terremoto. ore 16,49 del 18 gennaio 2017 una valanga maledetta si abbatte sull'*hotel* Rigopiano, causando la morte di ventinove Il personale della struttura e gli ospiti, tra cui quattro bambini, si ritrovano improvvisamente sepolti sotto un muro di neve. Per alcuni di loro sarebbero potuti essere giorni di svago, di spensieratezza, per altri ancora ordinari giorni di lavoro. E invece no. Seguono ore interminabili di angoscia, di speranza, di preghiera, che tengono l'Abruzzo e l'Italia intera con il fiato sospeso. Solo nelle prime ore del giorno successivo i soccorritori riescono a raggiungere il lungo del disastro con gli sci, perché le strade erano completamente bloccate dalla neve. Iniziano quindi le ricerche frenetiche, seguite con apprensione da tutti gli italiani, una corsa contro il tempo per salvare vite umane. Alla fine vengono estratte vive dalle macerie e dalla neve, purtroppo, solo nove persone, e tra queste i quattro bambini. In totale, undici sono i sopravvissuti: una tragedia immane, indimenticabile, alla quale anche il Presidente del Consiglio ha voluto tributare un ricordo incontrando lo scorso marzo i familiari delle vittime. In questi giorni, poi, è alle ultime battute il processo di appello e affido la mia fiducia alla giustizia per far luce su ciò che è accaduto, che si accertino le responsabilità. Oggi, come ogni anno da sette anni a questa parte, si svolgono proprio in queste ore le commemorazioni ufficiali a Rigopiano e anche noi, qui dall'Aula del Senato, vogliamo rendere omaggio al ricordo delle ventinove vittime e stringerci al dolore delle loro famiglie.

Senato, in sede di discussione del disegno di legge recante "Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione", ed altri. -*** ***Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, in materia di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni a statuto ordinario***

La seduta è tolta